L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Una delle qualità rivendicate da questa riforma di legge è proprio quella di riportare chiarezza sul riequilibrio tra l'Esecutivo e il Parlamento. Ebbene, l'emendamento 18.1 nasce da una

che nel periodo considerato il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri». Quindi, il peso dei provvedimenti di iniziativa

finanze*. Esprimo parere contrario per l'ovvio motivo che, scritto in questo modo, l'emendamento in discussione mira a creare una sorta di riserva indiana per i testi di iniziativa parlamentare

le ovvie ragioni di dinamica dei lavori dell'Aula, il voto elettronico. Non posso però ritirarlo perché non condivido il giudizio del Vice Ministro, dal momento che la riserva indiana ha consentito a suo tempo agli indiani di sopravvivere.

Si tratta forse dell'unico emendamento che presenta una qualche difficoltà di interpretazione sotto il profilo strettamente tecnico. Il testo al nostro esame ridefinisce in termini che complessivamente si possono anche condividere - a mio avviso - la distinzione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, spese determinate da fattore legislativo e spese discrezionali; insomma un qualcosa particolarmente complicato, da sempre oggetto di sforzi di comprensione da parte dei non addetti ai lavori; sforzi che, solitamente, vengono delusi. Qui però, attraverso il testo che giunge dalla Camera, modificativo del testo del Senato a proposito dei commi 4, 5 e 6, 6, abbiamo un effetto immediato, che non condivido, sul problema molto delicato - che segnalo alla Presidenza - che riguarda l'emendabilità ad iniziativa del Parlamento dei testi di dei testi di legge, in particolare della legge di stabilità e del bilancio. Si dice che le spese non rimodulabili sono quelle di cui l'amministrazione attraverso attività amministrative non ha un immediato controllo e, alla fine, si prevede che su questa componente della spesa

preferibile tornare al testo così com'era stato approvato in prima lettura dal Senato Peraltro, mi auguro che, come è accaduto questa mattina, ove quest'emendamento venisse respinto, in sede di applicazione della norma ci si comporti come se sostanzialmente il testo fosse rimasto quello approvato dal Senato.

impegnativo l'ordine del giorno che fra un po' illustrerò. Anzi, preannuncio

dell'Aula del Senato perché così si era espresso in prima lettura. Per quel che riguarda l'emendamento 21.2, anch'io credo che il Governo possa in un certo senso impegnarsi, nell'esecuzione di questi principi, a riportarsi a quanto più o meno era stato in precedenza previsto. Questo è però un impegno che può assumere il Governo.

Signora Presidente, non ho difficoltà ad assumere l'impegno testé lumeggiato dal senatore Morando, anche per un motivo molto semplice, perché in questo articolo noi passiamo ad una diversa classificazione delle spese,

richiederà un qualche tempo, durante il quale evidentemente si potranno anche fare i necessari aggiustamenti. Non dimentichiamo infatti che questa legge non si applica *d'emblée*, domani, dal 1° gennaio. Parte una procedura per cui alcune cose si applicano subito, altre richiedono un lavoro di cesello che postulerà il necessario apporto di tutte le forze presenti in Parlamento per arrivare ad una definizione finale. Quindi, anche in quella sede, nell'esame dei decreti delegati, l'apporto

a meno che evidentemente il dato non sia lapalissiano. Ovviamente questo dato viene poi confermato o meno con la controprova. Per nostra tranquillità, tanto perché, per esempio, in questa fase mi trovavo nel banco delle opposizioni,

La Presidenza ha cercato di richiamare l'attenzione di tutti quanti da circa 10 minuti sulla situazione ingestibile dell'Aula. Spero, per quel poco che rimane di questo provvedimento, di poter contare anche sulla sua collaborazione. Metto ai voti

considerata altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa;

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni;

con riferimento alla determinazione del conseguimento dell'obiettivo, cioè il passaggio al bilancio di cassa abbandonando il principio della competenza giuridica. In secondo luogo, sempre a mio avviso, sono stati eccessivamente allungati i tempi

lunga. Vorrei infatti fosse chiaro che sono consapevole della svolta radicale che, attraverso questa ipotesi, noi realizziamo rispetto alla normale decisione di bilancio e alla struttura del bilancio

- è l'unico Paese a caratterizzare la propria decisione di bilancio sostanzialmente secondo i principi della competenza giuridica. In tutti gli altri campi il principio della competenza economica, del bilancio di cassa, è stato affermato.

Ora, cari colleghi, capisco che questo può sembrare un tecnicismo, ma è un errore molto, grave perché tutta la logica che presiede al passaggio al bilancio di cassa è ispirata al tentativo di introdurre il principio di responsabilità nella verifica circa il conseguimento dei risultati ipotizzati. Se invece manteniamo di fatto, come il testo della Camera propone, il controllo preventivo sull'attività di gestione ad opera del dirigente della pubblica amministrazione, depotenziamo enormemente la portata straordinaria del passaggio al bilancio di cassa. in buona sostanza qual è la logica del dirigente pubblico: se può avere un bel parere preventivo sulla sua attività e poi mettersi tranquillo, a prescindere dai risultati, naturalmente sarà l'uomo più felice del mondo. Ora, vorremmo rendere un po' meno felici i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, soprattutto da questo punto di vista: basta con i controlli preventivi, introduciamo dei controlli sui risultati conseguiti. Si fa così dovunque la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere delle scelte che fa e dell'uso delle risorse che le si danno da gestire in un rapporto diretto dei dirigenti con il Governo, cioè con la struttura politica,

Per quanto riguarda l'idea di abbandonare i controlli preventivi, mi rendo conto della fascinosità del tema,

che consideriamo non certo una priorità ma almeno una necessità non più rinviabile se essa sarà realmente declinata nel quadro degli obblighi e dei vincoli europei e più in prospettiva del federalismo fiscale. Votiamo a favore così come abbiamo votato a favore la legge di riforma di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, perché riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di riforme istituzionali e strutturali, indilazionabili, alcune di queste a costo zero, che vanno avviate con urgenza perché i risultati che esse produrranno saranno apprezzabili soltanto in tempi medio lunghi. Votando no avremmo potuto fare una opposizione certamente più facile nel proporre sempre qualcosa di più e di meglio. Abbiamo invece scelto la strada responsabile nell'accettare le modifiche introdotte per evitare almeno che venisse approvata una legge centralista, ridondante e sbilanciata sull'Esecutivo. Sappiamo altrettanto bene che dobbiamo vigilare

si delinea una riforma che per alcuni temi, non certo marginali, è affidata alla legislazione delegata mediante la previsione di ben quattro diverse disposizioni di delega: dalle procedure di spesa in conto capitale al completamento della riforma del sistema dei controlli. Detto questo, farò alcune considerazioni che aiuteranno a comprendere meglio le nostre ragioni, mettendo un po' da parte il tecnicismo di questo disegno di legge e le specifiche competenze economiche che pure sono sempre utili per una valutazione politica più completa e approfondita. Anche perché, ascoltando le diverse posizioni espresse dai vari Gruppi nei

dato che io non mi iscrivo nella categoria dei bilancisti, non avendo alcuna competenza in tal senso. Laurence Peter diceva: «L'economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono accadute oggi». Questo anche per giustificare le diverse posizioni che all'interno dello stesso Gruppo sono maturate su questa riforma di contabilità. Resta il fatto - com'è stato ricordato, signora Presidente - che sono passati 31 anni dalla nascita della vecchia legge quadro n. 468 del 1978, e quindi saranno altre le valutazioni per le quali vedremo se questa nuova legge sarà stata in grado di innovare, non solo nella forma e nelle scadenze, ma piuttosto nel merito dei problemi di cui stiamo parlando. Per ora il nostro primo obiettivo è quello di dover uscire da un corto circuito istituzionale e politico, del quale questo centrodestra che ha governato il Paese per 8 anni sugli ultimi 15 deve sentirsi in parte o in buona parte responsabile. Da tempo la finanziaria, ridotta a una raccolta di centinaia di commi, aveva perso il suo ruolo centrale nell'impostazione delle manovre sui conti pubblici, diventando sempre meno occasione di discussione parlamentare e facendo sempre più un ricorso ai voti di fiducia. Poi da un paio di anni la finanziaria è stata resa scheletrica e ha lasciato il passo a decreti-legge che di fatto hanno ulteriormente usurpato e mortificato il ruolo del Parlamento nell'intervenire sui conti dello Stato, determinando nella sostanza una sorta di superamento dei vincoli che la Costituzione pone al bilancio. Questa dunque è la situazione di partenza.

la prima è avere qualcosa da dire; la seconda è dirla in modo adeguato e coerente al mezzo utilizzato, altrimenti si fa solo confusione o, peggio ancora, si fa propaganda. Oggi, a riforma approvata dopo il voto, abbiamo fornito un mezzo al Parlamento e a questa maggioranza, che ha la responsabilità di governare, spetta il dovere di mettere in campo idee, progetti e riforme. Nessuno di noi dell'Italia dei Valori ha mai pensato che l'idea geniale di Tremonti di una finanziaria leggera fosse risolutiva dell'assalto alla diligenza. Lo stiamo vedendo, e lo vedremo anche nei prossimi giorni, con la finanziaria che tornerà al Senato che risucchia il trattamento di fine rapporto, prosciuga la ricerca, fa tanti altri tagli, ma si scopre poi di manica larga per le somme stanziate a scatola vuota, con appositi commi al maxiemendamento, il cui contenuto sarà definito grazie a segnalazioni discrezionali, ad associazioni amiche, ai soliti enti finalizzati per lo sviluppo territoriale e a ONLUS, per una somma messa a disposizione di 520 milioni di euro. Nessuno di noi pensa che sia sufficiente cambiare un nome (da Documento di programmazione economico-finanziaria a Decisione di finanza pubblica) per recuperare il ruolo ormai del tutto trascurabile svolto dal Parlamento nella produzione legislativa recante oneri finanziari. Ce lo ha ricordato - come ho anticipato in discussione - un recente studio del Servizio bilancio del Senato, secondo cui nei primi otto mesi del 2009 il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri: in soldoni, su circa 14,6 miliardi di spesa per l'anno 2009, i finanziamenti decisi da Camera e Senato sono stati pari a 410.000 euro. Da sindaco di un piccolo straordinario Comune qual ero riuscivo a governare e a gestire maggiori risorse. Nessuno di noi Nessuno di noi dell'Italia dei Valori pensa che una Commissione per la trasparenza dei conti pubblici in più o in meno possa risolvere il problema della spesa pubblica. L'attuale Governo ha già trovato modo di mandare a casa la Commissione tecnica per la finanza pubblica che era stata precedentemente istituita a ha messo in un cassetto il suo rapporto elaborato sulla revisione della spesa pubblica, con il risultato - e questo lo dico al presidente presidente Baldassarri - che il Paese, nonostante l'assenza di importanti interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria simile a quanto si era già registrato nel precedente quinquennio del Governo Berlusconi 2001-2006. Nessuno dell'Italia dei Valori pensa che il contenuto del comma 6 dell'articolo 9, abolito alla Camera, avrebbe risolto il problema dell'alleggerimento del Patto di stabilità, se non si ha poi il coraggio di scelte più concrete per venire incontro alle esigenze degli enti locali. Infatti, proprio quando c'è bisogno di rilanciare l'economia attraverso gli investimenti i Comuni non possono spendere. Nei primi otto mesi del 2009 si sono persi per strada 2.150 bandi per opere pubbliche dei Comuni. Signora Presidente, senza riforme, il giorno in cui la crisi finirà e riprenderemo a crescere dell'1 per cento l'anno, come ci è stato detto, la disoccupazione rimarrà elevata per oltre un decennio. Il Governo ha i numeri necessari per portare a termine riforme importanti per l'emergenza e soprattutto per il dopo emergenza. Le scuse Le scuse che ancora in questi giorni si sentono circolare lasciano il tempo che trovano. Serve al Paese una politica straordinaria, capace non di vivere alla giornata del piccolo cabotaggio, dell'andamento dei sondaggi, dei colpi di scena, dei posti fissi e dei tagli IRAP, che servono a riempire le pagine dei giornali, ma capace di allungare lo sguardo e, nel tempo rimasto libero tra un lodo Alfano e un processo breve, di suscitare la speranza sui veri interessi del nostro Paese.

funzionali all'adozione dei documenti di programmazione finanziaria e anche i documenti contabili e finanziari su cui si regge il nostro Stato siano semplificati, efficienti, più accessibili e quant'altro,

un maggiore sforzo da parte dello Stato centrale nell'armonizzazione dei bilanci e soprattutto nella conoscenza di quale sia realmente, in maniera diretta e indiretta, il costo della finanza pubblica per il cittadino italiano.

Rispetto a ciò, è politicamente centrale in questo ragionamento che la relazione tra l'Unione europea e lo Stato italiano non sia intergovernativa, perché non è e non sarà più

sintonia e sinergia, soprattutto quando le decisioni del Parlamento europeo e la legislazione europea impegnino finanziariamente le finanze dello Stato e del sistema allargato della contabilità pubblica che riguarda le Regioni e il sistema delle autonomie locali.

di un controllo sulla trasparenza dei conti pubblici, sulla loro accessibilità e veridicità è stata declassata a Commissione con compiti meramente e blandamente conoscitivi. Tuttavia, la struttura di supporto tecnico, di cui parlava prima il collega Morando, è necessaria perché è lo strumento che consente di verificare l'andamento e l'efficienza del sistema della nostra contabilità pubblica. Quest'ultima non si fonda più su un unico soggetto centrale e protagonista, ossia lo Stato, ma vi è una polverizzazione di soggetti con pari dignità anche dal punto di vista del sistema della gestione delle entrate

dei controlli oggettivi del Parlamento, per mettere tutti nelle condizioni di conoscere qual è realmente lo stato della finanza pubblica allargata,

infatti evidente che se un Esecutivo vuole portare a compimento un programma di Governo, esso deve avere la forza e gli strumenti necessari per poterlo fare senza essere bloccato dal Parlamento.

nella legge di delega sul federalismo fiscale (quando le competenze in materia di controllo della fiscalità sono state attribuite

in qualche modo anche compiaciuti del fatto che si arrivi a fine anno alla loro approvazione. *(LNP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice ministro Vegas, vorrei esprimere il mio apprezzamento e quello del Gruppo della Lega Nord di legge n. 1937 riguardante la proposta di riforma della legge di contabilità dello Stato, che oggi ci accingiamo a votare. Esso rappresenta un importante passo avanti nel processo di aggiornamento e adeguamento, in chiave unitaria, del governo della finanza pubblica. Il presente disegno di legge consente il superamento di incertezze e di incoerenze nelle norme vigenti, mentre è in sintonia con il federalismo fiscale, con la necessità di contenere il disavanzo pubblico tramite un efficace ed efficiente impiego delle risorse con i vincoli imposti al bilancio pubblico dal Patto di stabilità e crescita. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge che ritengo meritevoli di considerazione. L'estensione delle regole di contabilità dello Stato alle pubbliche amministrazioni ristabilisce il principio di unitarietà del sistema economico della Repubblica, sancito dalla Costituzione all'articolo 117, ma che oggi si presenta frammentato e diversificato (ad esempio, nella sanità, coesistono sistemi contabili per cui al sistema delle rilevazioni di Stato si affiancano anche sistemi di natura economica; mentre in altri enti pubblici vengono adottati sistemi misti di natura economica e finanziaria). Tale principio, inserito nella delega al Governo, porterà alla convergenza dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni (così come definite dall'ISTAT all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge). La necessità della convergenza era emersa anche con la ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992, ma non ha ancora trovato compimento in Italia. Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche comporterà alcuni importanti cambiamenti all'interno delle stesse amministrazioni, quali, ad esempio, l'adozione di un piano di conti integrato, di comuni schemi di bilancio (articolati in missioni e programmi) e di principi contabili uniformi. L'armonizzazione consentirà un più facile consolidamento un più facile consolidamento nei bilanci degli enti controllanti (Regioni, Comuni e così via) dei bilanci delle aziende da esse controllate e un puntuale monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione. Probabilmente tale passo non sarà indolore per molti amministratori pubblici e per coloro che operano nel settore della contabilità; forse ci saranno resistenze da superare e conoscenze da approfondire. Tuttavia, la centralità di questa norma richiede che siano intrapresi in parallelo tutti gli sforzi possibili per superare i sistemi contabili attualmente in uso, anche in vista dell'attuazione di uno stabile federalismo fiscale. L'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili consentirà di integrare ed omogeneizzare i sistemi di controllo già applicati nelle varie amministrazioni pubbliche, con un risvolto positivo sulla loro efficacia. Un altro vantaggio sarà la condivisione in tempo reale, tra tutte le amministrazioni, delle informazioni finanziarie ed economiche. Da sottolineare che questa armonizzazione dei sistemi contabili è coerente e collegata con un pilastro fondamentale del federalismo fiscale che sono i costi standard. Altro aspetto è la riclassificazione del bilancio per programmi e missioni. Il bilancio dello Stato viene riclassificato in programmi e missioni e scompaiono i capitoli di spesa. I programmi diverranno le nuove unità di voto parlamentare, cioè «l'attenzione del Parlamento si focalizza sulle finalità delle spese e non sulle strutture che le gestiscono». Si prevede la scomparsa del capitolo di spesa, quale unità gestionale del bilancio. II Parlamento voterà per «aggregati omogenei di attività finalizzate al perseguimento di obiettivi individuati con le missioni», e non più per unità previsionali di base. Il bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche diventerà più flessibile per l'effetto sinergico dell'adozione dei programmi quali unità di voto e della possibilità di effettuare rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all'interno delle missioni inserite in ciascun programma; la flessibilità è "con alcuni limiti riguardanti le sole spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti" La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità, titolare dei risultati raggiunti, con indubbi risvolti positivi in termini di recupero del controllo sulla spesa e della misurabilità delle prestazioni. Dall'approvazione di questo disegno di legge deriverà l'opportunità di adottare un sistema per la valutazione dei risultati, dei processi e dell'impiego delle risorse attuato dalle pubbliche amministrazioni; il tutto comporterà vantaggi in termini sia di conoscibilità dei fatti di gestione che di trasparenza. La riclassificazione delle poste per missione è già stata introdotta nella legge finanziaria con l'indicazione del programma a cui si riferisce. I nuovi strumenti di programmazione e l'ampliamento dell'orizzonte temporale di loro applicazione garantiranno una maggiore certezza

L'orizzonte temporale triennale si ripresenta all'interno dei documenti programmatici e contabili dello Stato. Il nuovo documento di programmazione «Decisione quadro di finanza pubblica» (DQFP) definisce infatti per un triennio, in sostituzione del DPEF, il livello complessivo della spesa triennale dello Stato e gli obiettivi di ciascun livello di decisione. II disegno di legge in esame modifica la struttura del bilancio dello Stato (sia annuale che pluriennale), che risulta rafforzato quale strumento di allocazione e gestione delle risorse pubbliche. rende inoltre più snella la legge finanziaria in seguito alla soppressione degli interventi per lo sviluppo che concorrono ad aumentare le spese, all'accorpamento e alla riduzione del numero delle tabelle allegate (da sette a quattro), all'eliminazione dei suoi collegati e alla soppressione dell'obbligo di copertura degli oneri correnti. Questo è il punto delicato del disegno di legge, specialmente per la cultura italiana - diverso sarebbe nel Centro e nel Nord Europa - e nutro alcune perplessità riguardo a quest'ultimo aspetto, ovvero l'eliminazione degli attuali vincoli di copertura degli oneri correnti previsti per l'attuale legge finanziaria. Ciò consentirebbe la possibilità di adottare misure espansive attraverso la legge finanziaria entro il limite del saldo netto da finanziare, anche per le spese di natura corrente. concludo quindi preannunciando il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame, auspicando che lo stesso, dati gli importanti risvolti che avrà sulla futura vita dello Stato, possa trovare il massimo consenso tra le compagini politiche qui rappresentate.

il Gruppo del Partito Democratico del Senato non confermerà il voto favorevole al disegno di legge di riforma della legge di bilancio già espresso al termine della prima lettura presso questo ramo del Parlamento. Il nostro voto sarà di astensione. Ci troviamo di fronte a una vera novità: al Senato il testo esitato dal Comitato ristretto ottiene i voti favorevoli di tutta l'Aula (con l'eccezione del Gruppo dell'Italia dei Valori) alla Camera il provvedimento subisce incredibili e profonde modifiche che, se da una parte apportano alcuni piccoli miglioramenti, dall'altra peggiorano il testo, espungendo e decurtandolo di importanti e qualificanti parti approvate dalla quasi unanimità del Senato della Repubblica. Ripeto, signor Vice Ministro: dal Senato della Repubblica, non dal Comune di Coccaglio, giusto per farle un esempio. Il provvedimento è infine approvato in quella sede con i voti favorevoli di tutta l'Assemblea.

il diritto e il dovere di meglio legiferare per il bene del Paese (e questo noi stiamo cercando di fare). Nella nostra Costituzione, signor Vice Ministro, non è scritto da nessuna parte

lei ha detto le stesse parole alla Camera quando avete votato il testo modificato? Invece di ricordarci come abbiamo votato alla Camera, lei e il ministro Tremonti - che, mi permetto di ricordare, anche oggi ritiene non importante essere presente in quest'Aula, vista la scarsa rilevanza della legge che stiamo per approvare - dovreste trarre il dato politico che questo testo non è condiviso dal famoso legislatore nella sua interezza e che una legge di riforma così importante non si licenzia senza il consenso pieno e alto dei membri delle due Camere. Così facendo, signor Vice Ministro, si ripercorrono errori già commessi prima da noi, sul Titolo V della Costituzione, e poi da voi, in materia elettorale e con il lodo Alfano. Se l'obiettivo era quello di approvare il disegno di legge di riforma in tempi stretti, potevate ottenerlo a luglio, facendo confermare alla Camera il testo licenziato dal Senato, permettendo al Paese di affrontare la sessione finanziaria 2010 con la nuova legge di stabilità. Al contrario, alla Camera lo avete profondamente modificato, per alcuni versi peggiorandolo, e qui in Senato lo avete blindato, sia in Commissione bilancio che in Aula. Perché, colleghi della maggioranza - ancorché poco presenti in quest'Aula e molto distratti - non vi interrogate sul fatto che anche il vostro presidente della Commissione finanze, il senatore Baldassarri,

Il testo del Senato disegnava un profilo riformatore del quadro di contabilità pubblica del Paese e dei ruoli fra Governo e Parlamento. La riforma restituitaci azzera molti di questi profili riformatori. Con questo testo, che cosa consegnate al Paese? Una riforma con un bilancio dello Stato più semplificato? No, perché con questo testo il bilancio non diventa più chiaro ed accessibile ai cittadini. Volete consegnare una riforma dei ruoli di Governo e Parlamento nella gestione del bilancio pubblico? No, perché con questo testo il Governo conferma il proprio ruolo nella gestione del bilancio e al Parlamento vengono sottratti gli strumenti di autonoma lettura, di verifica e riscontro della contabilità pubblica.

è ridotta ad un mero strumento di controllo del deficit, è privata della sua natura di strumento di politica economica e svuotata dell'effettiva capacità di controllo da parte del Parlamento sull'operato del Governo. Quattro erano i punti qualificanti sui quali il Senato aveva bene operato in prima lettura, che costituivano la premessa per un'azione riformatrice e che alla Camera avete modificato in peggio: la trasparenza dei conti pubblici e il rapporto tra Governo e Parlamento, il Patto di stabilità interno, i vincoli sulla spesa e il passaggio al bilancio di cassa. Sulla trasparenza dei conti pubblici, tutti eravamo d'accordo, nel maggio scorso, sul fatto che il Parlamento è carente degli strumenti adeguati per farlo. La Commissione per la trasparenza dei conti pubblici e il Servizio unico del bilancio dovevano costituire la strumentazione di partenza, senza la quale il restante lavoro di riforma della legge di bilancio sarebbe stato inutile. La Commissione per la trasparenza avrebbe reso il Parlamento autonomo, rispetto al Governo, nel compito di verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica; con la struttura unica di bilancio, sarebbero stati forniti elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Entrambi questi articoli, il 4 e il 7, sono stati modificati o soppressi alla Camera. L'articolo 4 prevede ora un generico controllo parlamentare. Ma ragionate, colleghi della maggioranza, come può il Parlamento controllare autonomamente l'operato del Governo, se è il Governo stesso a fornire tutte le informazioni? Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, controllare i dati che il Governo trasmette, se il primo non conosce le metodologie attraverso le quali i dati sono stati calcolati? La struttura unica di controllo avrebbe rafforzato il potere del Parlamento sul Governo: perché la Camera l'ha soppressa, signor Vice Ministro? Perché un ramo del Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, ha ridotto la sua stessa capacità di controllo sull'operato del Governo? Sarebbe terribile scoprire, signor Vice Ministro, sull'operato del Governo? Sarebbe terribile scoprire, signor Vice Ministro, che le ragioni vadano individuate nella mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico. La soppressione del Servizio unico di bilancio sembra purtroppo dimostrare che la resistenza delle burocrazie coinvolte nella riforma sia più incisiva della stessa volontà politica di riforma: così facendo, quale azione riformatrice introduce il vostro Governo? Nessuna! Sul Patto di stabilità interno, colleghi della Lega, anche voi avete soppresso i commi 6 e 7 dell'articolo 9 (ora articolo 8): andatevi a rileggere quello che avete soppresso

di avere parametri per valutare i risultati raggiunti in termini di aggregati; il secondo - te lo ricordi, collega Vice Presidente della Commissione bilancio? - era quello di individuare le responsabilità nel caso di un eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Oggi lo avete abrogato con il voto alla Camera e lo licenziate in questo modo,

sono riusciti a controllare la spesa proprio in virtù della programmazione disaggregata in termini di entrate e di spese, oltre che per avere attribuito un tetto alla spesa. Il Senato introduceva nella lettera *g)* questa strumentazione solo a fini conoscitivi, eppure, pur non essendo vincolante, innovava nel nostro sistema contabile, portandolo verso un metodo di programmazione orientato all'individuazione di vincoli sulla spesa. Perché è stato tolto? Perché avete cancellato una parte della lettera *g)*,introdotta nell'attuale lettera che costituiva problemi? Perché avete soppresso la possibilità di verificare gli obiettivi del Governo disaggregati piuttosto che solo i saldi?

che una vera riforma. Citerò solo alcuni esempi: alla lettera *d)*, avete reintrodotto un sistema di controlli preventivi che il collega Morando ha ricordato essere stato eliminato nei primi anni '90;

qual è l'innovazione che il disegno di legge introduce in questa lettera? Quale il metodo di competenza più che di cassa che si rileva nella lettera *d)*? Nella lettera *h)*, ancora una volta enfatizzate una contabilità di competenza e non di cassa: con il testo approvato dalla Camera, che qui avete blindato, avete reintrodotto un approccio preventivo in materia di controllo, rovesciando la logica funzionale del controllo *ex post*, orientato alla verifica dei risultati, e scardinando il meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza come l'avevamo approvato in Senato. In conclusione, signora Presidente, il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera ha ridotto e sminuito la portata innovativa della riforma di contabilità così come approvata dal Senato: la trasparenza e l'indipendenza dell'informazione statistica non sono più garantite, ma diventano funzione del *commitment* politico, e al Parlamento non sono garantiti gli strumenti per il funzionamento indipendente del proprio ruolo di controllo e di indirizzo politico. Va dato merito alla Camera di aver perfezionato il raccordo tra il disegno di legge ed il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. tale miglioria, sommata alle ingiustificate soppressioni prima esplicitate, non ci consente di votare favorevolmente questo testo. Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico si asterrà. Rimane il compito affidato al Presidente del Senato, congiuntamente al Presidente della Camera, come più volte ripetuto dal Vice Ministro oggi, di avviare effettivamente e con l'estrema urgenza del caso la riforma dei Regolamenti parlamentari. si tratta di un passaggio divenuto ormai decisivo e non più eludibile per il buon funzionamento della legge che stiamo approvando. Il voto di astensione che oggi ci apprestiamo ad è un voto di rispetto per l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto prima e dall'Aula del Senato poi durante la prima lettura, ma è un voto di non condivisione di alcune sostanziali scelte sbagliate della Camera, che hanno soppresso e abrogato articoli e commi fondamentali approvati dal Senato, ed è, colleghi senatori, un voto di ferma protesta per la scelta operata dal Governo, che ha chiesto alla sua maggioranza di non operare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, privilegiando così la sintesi al ribasso, piuttosto che la bontà di un risultato di qualità per il futuro dei conti pubblici del nostro Paese.

FRATIN *(PdL)*. Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, senatrici e senatori, con il voto che l'Aula del Senato tra poco esprimerà in seconda lettura sul disegno di legge n. 1397 giunge a conclusione un ampio processo di revisione delle norme che regolano la contabilità e i rapporti tra i diversi livelli di finanza pubblica. Si tratta di un processo articolato che tuttavia ha permesso di raccogliere, almeno in fase di elaborazione, un'ampia adesione rispetto ad un'esigenza di riforma sentita e sollecitata da tutte le forze politiche e dai diversi Gruppi parlamentari. Il fatto che tale riforma attenga a un settore specifico dell'attività delle pubbliche amministrazioni non toglie nulla alla rilevanza del momento, che appare, a mio avviso, sottovalutata in seno all'opinione pubblica e al sistema dell'informazione, forse per la difficoltà di approccio vista la tecnicità della materia. Nondimeno occorre sottolineare che un cambiamento così profondo delle regole per la definizione dei meccanismi che presiedono alla formazione dei conti pubblici, nelle diverse fasi e con i diversi protagonisti istituzionali, acquista una particolare rilevanza proprio perché è stata in gran parte condivisa tra maggioranza e opposizione, nello spirito che quest'Aula ha formalmente stabilito nelle mozioni sulle riforme istituzionali approvate pochi giorni fa. Non mi addentro nei dettagli delle modificazioni introdotte alla proposta di legge nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Il testo che è tornato all'attenzione del Senato conserva in gran parte le sue caratteristiche, così come la *ratio* che lo aveva ispirato,

e rappresentano un utile miglioramento della qualità della normazione acquisita nel passaggio tra le Camere legislative. Altre hanno natura sostanziale e sono frutto di scelte in parte diverse rispetto a quelle compiute dal Senato in prima lettura. Voglio qui citare, a titolo di esempio, le modificazioni introdotte per la necessità di meglio coordinare il disegno di legge con la sopravvenuta legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale (legge n. In particolare, si introduce nella succitata legge una nuova disposizione, all'articolo 2, comma 1, relativa alla delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione delle autonomie territoriali. La nuova norma aggiunge alla delega la finalità di armonizzare i sistemi contabili, gli schemi di bilancio delle autonomie territoriali e i relativi termini di presentazione e approvazione in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Un'ulteriore innovazione, che è stata peraltro lungamente dibattuta e che non soddisfa certamente gran parte dei membri del Senato, è costituita membri del Senato, è costituita dalla soppressione dalla noma che prevedeva l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica. In tal modo la Camera In tal modo la Camera ha voluto ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito ordinario delle Commissioni bilancio, quindi sarà responsabilità di Senato e Camera trovare il nuovo percorso nell'ambito dei Regolamenti parlamentari. In tale quadro si deve ancora sottolineare l'eliminazione - purtroppo - della previsione (contenuta nell'originario l'articolo 7) mediante cui si stabiliva che gli elementi tecnici di supporto del controllo parlamentare sulla finanza pubblica consistessero in un'unica struttura tecnica da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere.

un rafforzamento anche del ruolo parlamentare nei confronti dell'Esecutivo. A fronte di tali innovazioni, resta sostanzialmente confermata l'adesione al metodo della programmazione per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa; rispetto alla normativa vigente, la disposizione in esame estende peraltro tale metodo alle previsioni di bilancio del complesso delle amministrazioni pubbliche. Il comma 2 dell'articolo 7, che reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, annovera, come voluto dalla Camera, anche il disegno di legge di assestamento, che il Governo dovrà presentare entro il 30 giugno di ogni anno. La nuova impostazione del ciclo di bilancio, già definita in prima lettura, è volta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni Con ciò arriviamo quindi al nodo centrale del disegno di legge all'esame, ovvero la rideterminazione della diversa struttura degli strumenti di finanza pubblica, anche riguardo al ciclo temporale in cui sono collocati finanziario. Tra gli aspetti positivi si deve ancora ricordare la triennalizzazione della manovra finanziaria, realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione, si formalizza e inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. che conteneva una serie di misure al fine di conseguire per ciascuno degli esercizi finanziari nel triennio 2009-2011 gli obiettivi programmatici discendenti dalla manovra definita con il DPEF. Sulla base della normativa in via di approvazione si vincola il Governo a proporre una manovra triennale, salva ovviamente la possibilità di introdurre cambiamenti di scelte politiche all'interno dell'impostazione della manovra così definita. Comunque, in linea generale, la scelta di rafforzare l'efficacia degli strumenti di programmazione economica, sancendo in modo più puntuale l'impostazione triennale della manovra di finanza pubblica, raccoglie anche le sollecitazioni dell'Unione europea a orientare la configurazione del quadro contabile di riferimento per la decisione di finanza pubblica in senso analogo alle esperienze di altri Paesi partner. In proposito si inserisce anche la valutazione che faceva in merito al bilancio di cassa come obiettivo il senatore Lusi nell'intervento che mi ha preceduto.

il Parlamento ha già varato la manovra finanziaria relativa all'anno in corso e quella, in corso di definizione, riguardante il 2010. Questo provvedimento rappresenta quindi, dopo le molte attese e auspici, la riforma della sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che il varo della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati comportasse un impegno legislativo tale da impegnare per mesi il lavoro delle Camere, anche a causa della prassi invalsa di utilizzare tali strumenti, in origine di natura programmatoria e finanziaria, per dare risposte a molteplici interessi categoriali, territoriali, afferenti a singoli tematiche e materie. In tale prospettiva il presente disegno di legge si configura come un grande passo verso una sistematizzazione, una formalizzazione stabile della decisione assunta all'avvio della legislatura dal Governo di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni.

si creano dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e di indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo e affinché, nel contempo, allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed efficace delle politiche e delle scelte realizzate dall'amministrazione, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare. Il vasto consenso, almeno nella fase dibattimentale, se non nel voto finale - purtroppo - per le annunciate astensioni, contribuirà a stimolare l'Esecutivo nell'esercizio delle deleghe che vengono ad esso conferite, in modo da consentire una piena operatività delle nuove regole contabili già dal prossimo anno finanziario. signora Presidente, con un ringraziamento al relatore Azzollini e a tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza che sia in prima lettura che in questa ultima fase hanno contribuito

non abbiano ricevuto da questa seduta grandi esempi di disciplina.

poiché ero e resto profondamente convinto che il testo del disegno di legge approvato dal Senato fosse estremamente coerente con il codice genetico del mio partito, il Popolo della Libertà, Popolo della Libertà, e con il programma del mio Governo, il Governo Berlusconi, e poiché sono convinto che il testo che ci è tornato dalla Camera abbia perso queste caratteristiche genetiche, come ho tentato di

Signora Presidente, intervengo soltanto per ringraziare, alla fine di questi lavori in terza lettura, tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito e che hanno proposto, ancora con grandissima competenza e con grandissima passione, le loro posizioni e le loro opinioni, indipendentemente, naturalmente, dall'espressione del voto, che sarà quella che ciascun Gruppo e ciascun senatore deciderà. Voglio ancora confermare

per alcuni versi profondamente dialettico, ma che ha visto comunque tutti i parlamentari profondamente coinvolti di una legge di sistema, speriamo destinata a durare a lungo, certamente suscettibile di miglioramenti e di approfondimenti, ma che viene portata a conclusione con il sicuro intento da parte di tutti di contribuire ad un miglioramento della dialettica fra Governo e Parlamento, ad una migliore funzione del Parlamento, in particolare nella materia delicata della finanza pubblica, e, soprattutto, alla ricerca di una normativa che vada nell'interesse del Paese.

ai colleghi dell'opposizione e ai colleghi della maggioranza tutti che si sono esercitati davvero, lo ribadisco, in una pagina del Parlamento che sicuramente fa onore al nostro Paese. Di ciò vi ringrazio di cuore tutti.

non di agevole lettura, comunque una riforma di struttura delle regole del gioco. Il fatto che il Parlamento, partendo in modo autonomo, riesca a definire le regole del gioco, che non riguardano solo il Parlamento ma l'intera struttura

Signora Presidente, signori senatori, sarò estremamente breve. Come tutti coloro che si occupano della materia sanno perfettamente, l'articolo 2947 del codice civile prevede che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni, come sappiamo tutti, se si tratta di fatto illecito e soli due anni se si tratta di un fatto che dipende dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

questa aggiunta all'articolo 2947 del codice civile si dà la stessa facoltà di procedere entro lo stesso termine di prescrizione anche all'imputato a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno,

presidente Berselli ha trovato il consenso unanime di tutta la Commissione.

Questo disegno di legge introduce appunto un principio di parità, naturalmente in presenza di un imputato cui giunga una sentenza di

Signora Presidente, onorevoli colleghi, quella al nostro esame è una norma che ha carattere assolutamente particolare e tuttavia la sua importanza, come i colleghi hanno detto, non è da sottovalutare. Si tratta, sostanzialmente, di riequilibrare ed omologare le facoltà in capo all'imputato e al responsabile civile rispetto alle facoltà che già sussistono in capo alle proprie controparti.

o il responsabile civile che non si fosse premurato di mettere in atto atti interruttivi veda ormai prescritto il suo diritto. Si verifica spesso, particolarmente in talune fattispecie di reato, ad esempio in quelle che attengono alla diffamazione, alla calunnia, ed altre ancora, ma specificamente in questa famiglia di reati, che invece l'imputato ed il responsabile civile abbiano una naturale e legittima aspettativa di carattere risarcitorio,

con un'interpretazione estensiva della stessa norma taluni hanno ritenuto che già vi fosse inclusa tale facoltà, si è ritenuto invece che si dovesse esplicitamente sancire questo diritto in capo all'imputato e al responsabile civile. La *ratio* è dunque giuridicamente assolutamente condivisibile e, non a caso, è stata condivisa da tutti i settori della Commissione, e oggi dell'Aula. Pertanto,

come il disegno di legge presentato dal presidente Berselli, ma sottoscritto - cosa assai positiva - dai rappresentanti di tutti

la disciplina costituzionale del giusto processo. Oggi dalla disciplina attualmente prevista dall'articolo 2947 del codice civile origina una disparità di trattamento - come è già stato sottolineato - a danno dell'imputato che non sia parte la sua azione risarcitoria nei confronti del querelante o di chi si sia costituito parte civile si prescrive a decorrere dalla data data della denuncia-querela e non - come invece si prevede nel disegno di legge in esame - dalla data della sentenza definitiva di assoluzione, mentre è certamente giustificata la diffusa ricorrenza comportamentale comportamentale che vede l'imputato promuovere l'azione di risarcimento soltanto quando il procedimento penale a suo carico si sia definitivamente concluso con l'assoluzione. La tutela di chi ha ragione è lo scopo principale di questo provvedimento. Penso ad esempio a chi sia stato ingiustificatamente calunniato: costui oggi viene onerato non soltanto della difesa nel processo penale, non solo dell'azione nel processo civile, ma anche della irragionevole durata dell'uno e dell'altro. L'opportunità dell'equiparazione si pone in termini anche sostanziali. L'iniquità della differenza tra i diversi termini di decorrenza pesa anche a causa della lunga durata dell'accertamento giudiziale, perché se tale accertamento avvenisse in termini solleciti i due diversi tempi di decorrenza, quello oggi vigente e quello che si intende introdurre, si collocherebbero ad assai più breve distanza e non accadrebbe che i diritti di chi risultato essere infine il vero danneggiato risultino quasi sempre largamente prescritti. Il dettato costituzionale del giusto processo vuole anche che la durata del suo la durata del suo svolgimento non rechi pregiudizio a chi ha ragione. L'approvazione di questo progetto non è pertanto solo auspicabile per ragioni di buonsenso, come recita la relazione al testo inizialmente introdotto, ma anche e soprattutto per ragioni di giustizia sostanziale.

Signora Presidente, intervengo brevemente in dichiarazione di voto sull'emendamento. Si tratta di una questione tecnica che si limita ad aggiungere l'aggettivo "irrevocabile"

Signora Presidente, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori sarà favorevole al provvedimento in esame. Già in Commissione il rappresentante dell'Italia dei Valori aveva dato il suo assenso. Voglio ricordare che stiamo parlando della prescrizione dell'azione risarcitoria derivante da un fatto considerato dalla legge come reato. Il nostro legislatore, nel prevedere l'istituto giuridico della prescrizione, ha voluto intendere che ogni diritto si estingue, se non esercitato entro un determinato periodo di tempo da parte del legittimo titolare. Quindi Quindi si è cercato di evitare che l'inerzia del titolare del diritto esercitabile possa essere prolungata oltre un limite ragionevole.

mentre la persona offesa del reato, la parte civile, poteva esercitare l'azione risarcitoria in un certo tempo, per l'imputato assolto con sentenza passata in giudicato o irrevocabile si prevedeva irrevocabile si prevedeva che il diritto ad esercitare l'eventuale azione risarcitoria decorresse dal momento della presentazione della querela e non dal momento in cui la sentenza fosse passata in giudicato e quindi fosse stato acclarato in modo definitivo che l'imputato era stato assolto. Ovviamente si richiede che la persona offesa versi in colpa grave, quindi che vi sia stata una denuncia

ingiusta ha conseguenze gravi e dannose per chi la subisce. E' una lesione ai diritti del proprio vivere, all'immagine, all'onore, alla reputazione e quindi è corretto che, nell'ipotesi in cui un imputato esca assolto da un procedimento penale, possa, nelle condizioni indicate dall'articolo 2947 del codice civile, esercitare anch'egli l'azione risarcitoria. Credo che questa lacuna andasse colmata, per cui l'Italia dei Valori voterà favorevolmente a questo provvedimento.

la quale fin dal primo momento ci siamo resi disponibili per una rapida approvazione sia in Commissione che in Aula. Si tratta di un provvedimento che non solo pone fine ad una

L'aver ripreso un binario corretto, con la tutela eguale di tutti i soggetti che possano trovarsi in determinate condizioni (in modo particolare l'imputato che venga assolto con sentenza irrevocabile di assoluzione), consente sostanzialmente di enfatizzare anche un'altra circostanza. Anche nel processo

Signora Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge al nostro esame, che è stato sottoscritto, come prima ha ricordato il Sottosegretario, dai Capigruppo in Commissione giustizia di tutti i movimenti rappresentati in Senato. Si tratta di un intervento - come è già stato sottolineato - di carattere ortopedico sul codice civile, finalizzato a chiarire meglio il momento di decorrenza della prescrizione del risarcimento del danno in una fattispecie specifica.

in esame, che avevamo già avuto modo di esplicitare nei lavori di Commissione. Non potrebbe essere altrimenti, perché esso è stato sottoscritto anche dal Capogruppo

sposta sostanzialmente rispetto al processo la posizione di chi si vede ampliati i termini per poter esercitare un'azione risarcitoria,

Presidente, in telegrafica sintesi, anche perché i contenuti sono già stati ampiamente illustrati, vorrei sottolineare che non si tratta semplicemente di una norma di buon senso ma, viceversa, di un passaggio tutt'altro che trascurabile, avuto riguardo a un profilo di giustizia sostanziale. Dobbiamo ringraziare il Presidente e gli altri Capigruppo che hanno ritenuto di convergere

il diritto al risarcimento del danno laddove si sia stati oggetto di un'accusa ingiustificata. Viene così sanata un'aporia di sistema

Siamo intervenuti, questa aporia è stata sanata e si è tra l'altro evitato che si potesse arrivare a un contrasto di giudicati, sussistendo più quella pregiudiziale penale vigente nel preesistente codice e quindi la possibilità di introdurre azioni civili in contemporanea rispetto al processo penale. È un lavoro che la Commissione ha svolto all'unisono e credo che, da questo punto di vista, non si possa che essere ampiamente soddisfatti del risultato raggiunto. È con l'auspicio che si possa procedere introducendo altri tasselli fondamentali per il giusto processo, che prevede necessariamente un'assoluta parità di trattamento e di posizione fra le varie parti processuali, che il Gruppo del Popolo della Libertà esprimerà il proprio voto favorevole.

colleghi, il disegno di legge n. 1929, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni,

di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, dà seguito all'impegno assunto dal Governo, su sollecitazione parlamentare, di annullare il concorso riservato per dirigenti scolastici dell'anno 2004 per la Regione Sicilia signor Sottosegretario, che questo sia il primo di una lunga serie di ricorsi di altre Regioni dei quali ci dovremo occupare in tempi più o meno brevi), laddove, a seguito di un ricorso da parte di alcuni concorrenti dichiarati non idonei, che lamentavano illegittimità procedurali quanto alla composizione della commissione, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia dichiarava nulli gli atti in base al principio del collegio perfetto. Le conseguenze di questo annullamento le pagano i docenti che - a mio avviso - sono sono i meno responsabili, perché le maggiori responsabilità appartengono a chi ha gestito il concorso e che ha mancato di controllare eventuali illegittimità degli atti concorsuali. Con il provvedimento al nostro esame, mentre si annullano le procedure concorsuali, si dispone che i dirigenti che erano stati dichiarati vincitori e che avevano assunto l'incarico rimangano nelle rispettive sedi sino all'espletamento del nuovo concorso, che si auspica avvenga in tempi rapidi, anche al fine di non ingenerare dubbi di legittimità sugli atti adottati nell'esercizio delle funzioni e di assicurare il corretto svolgimento dell'anno scolastico.

prevede giustamente l'annullamento del concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, come peraltro era previsto da un emendamento soppressivo che, di quel provvedimento, fu presentato sia dal sottoscritto, a nome del Partito Democratico, sia dal senatore Giambrone, a nome dell'Italia dei Valori, e che fu inspiegabilmente bocciato dalla maggioranza.

atti disciplinari e didattici - pensate a presidenze di collegi docenti - e a decisioni prese

«Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma». In realtà, in questo provvedimento il Governo si fa carico anche del tema della continuità didattica

magari incauta - nel precedente provvedimento salva-precari (che riguardava «solamente» 28.000 insegnanti incaricati annualmente)

i cui figli frequentavano la scuola elementare ha cambiato gli insegnanti con la riforma del modulo, passando all'insegnante unico.

Vi è però una preoccupazione di serietà (mi rivolgo in proposito al sottosegretario Pizza, che è sempre presente anche in Commissione),

nuovo concorso venga svolto entro il 31 agosto, perché queste persone non hanno colpa per l'invalidazione del loro concorso: la colpa è altrove, lo sappiamo.

che cercava di rimediare in qualche modo all'annullamento del concorso. In altre parole, si cercava di creare una soluzione legislativa per non ottemperare a una precisa sentenza che chiedeva

Questo avremmo dovuto fare e invece non lo abbiamo fatto. Ricordo ai colleghi, a quei pochi che seguono questo dibattito, la Commissione affari costituzionali (e, se non vado errata, anche la Commissione giustizia) aveva segnalato l'irregolarità di quel comma a quest'Aula,

Rusconi, chi oggi ha preso in mano una scuola da tre mesi non può essere sostituito con incarichi provvisori, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista del funzionamento scolastico),

Mi riferisco alla seguente formulazione: «(...) il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto». Se non accogliamo o non abbiamo altre assicurazioni sull'emendamento 1.2 che abbiamo proposto, che fissa una data,

di un concorso annullato. Voglio ricordare a tutti voi - anche se lo sapete perfettamente - che nella pubblica amministrazione la sede assegnata corrisponde ad un punteggio ottenuto proprio in quel concorso che dà diritto all'opzione di scelta.

I risultati del concorso sono indifferenti alla possibilità di scelta della

almeno la modestia di riconoscere i vostri errori! Non l'ho mica fatto io questo decreto, siete stati costretti a farlo voi!

Presidente, in appena due mesi, come è stato ricordato, riaffrontiamo un argomento per il quale oggi c'è una conoscenza ed una responsabilità che pesa sul Parlamento.

ha interamente riformato il giudizio di primo grado, decidendo di annullare il concorso per dirigenti scolastici, bandito il 22 novembre 2004 per la selezione regionale.

Eppure in questi organismi ci sono giudici togati. Forse non è un buon esempio di gestione della giustizia! Non escludo che questa decisione del Consiglio superiore possa essere frutto di

poiché nell'isola c'è stata uniformità alla legge e al bando come in tutta Italia. Oggi siamo in presenza di una ulteriore sentenza di ottemperanza alla quale il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia dovrà dare seguito entro il 12 gennaio 2010. Ciò significa che 427 presidi che hanno espletato un concorso - vincendolo non avranno più la qualifica di dirigenti scolastici. La proposta del Governo ci mette una pezza, tuttavia questi presidi saranno retrocessi a semplici incaricati, perdendo comunque autorità ed entusiasmo, nonché il rispetto dei loro sottoposti. Questa realtà porterà le 427 scuole siciliane nel caos,

Forse non sarebbe stato opportuno mantenere per quindici anni un presidente del CGA che, tra l'altro, ha prodotto ricorso alla Corte costituzionale affinché venisse soppresso l'organismo che lui stesso presiedeva. È pensabile che si possa procedere all'esame di un ricorso senza averlo notificato almeno ad uno dei controinteressati? Il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione - come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - prevede che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti. Non si è tenuto conto della imprevedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente alla impugnazione degli atti inerenti la procedura, stante che la stessa è stata rinnovata. Ma cosa porta a questa sentenza? La nomina di sottocommissioni imperfette. Eppure è la legge e il conseguente bando che prevede un unico presidente del concorso e la nomina di due componenti per ogni sottocommissione. Nei fatti la direzione generale dell'ufficio scolastico per la Sicilia si è uniformata alla direttiva ministeriale n. 1160 del 19 maggio 2005, impartita dal Ministro dell'istruzione. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che l'appello amministrativo regionale è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo insufficiente la motivazione. La pubblicazione della graduatoria rende vano l'appello nel caso in cui non fosse garantito il contraddittorio tra tutti i vincitori attraverso l'impugnazione della graduatoria definitiva. I graduati favorevolmente non possono essere incisi dall'esito di un giudizio dal quale sono rimasti assolutamente estranei. I verbali della sottocommissione del concorso costituiscono atto pubblico che, pertanto, fa fede fino a querela per falso. Non risulta che nessuno dei ricorrenti abbia proposto tale querela. Nei prossimi giorni la direzione scolastica regionale dovrà procedere al licenziamento dei presidi, anche se questa legge in discussione consente di lasciarli nelle loro sedi come incaricati. legali per adire il giudice del lavoro, poiché viene meno un contratto definitivo stipulato tre anni fa e regolarmente osservato nell'espletamento delle loro funzioni. Nel contempo, non mancheranno di chiedere al Ministero competente il risarcimento dei danni derivanti da una decina di motivazioni, per le quali non sarà facile sostenere che non sono dalla parte della ragione. Tra i presidi vincitori di questo concorso ci sono anche coloro i quali, pur avendo diritto, non parteciparono al concorso riservato poiché avevano vinto quello ordinario. Questi presidi, se retrocessi, dovrebbero ritornare nei posti originari che già sono stati occupati da altri, che di conseguenza resterebbero senza posto. Mi auguro che non si verificheranno altre vicende come quella dei dirigenti scolastici siciliani, che ha causato non poco disgusto tra la popolazione. Forse dopo questa sentenza tanti altri si sentiranno incoraggiati a percorrere lo stesso *iter*, vanificando anche lo sforzo messo in atto per la selezione dei pubblici dipendenti. Colgo con interesse lo sforzo del Governo nella ricerca di una difficile soluzione. Sono fiducioso che si farà il possibile per ridare serenità alla scuola siciliana, che oggi è minata da forti preoccupazioni. Può essere opinabile quanto si vuole, ma al punto dove siamo è imprescindibile avviarsi verso un corso-concorso, di breve durata, per chiudere speditamente questa non edificante realtà. È nell'interesse generale ridare fiducia alla scuola siciliana e ai suoi dirigenti scolastici; pertanto si impone una decisione sollecita e condivisa. Questa situazione dei presidi, che mette a soqquadro l'intero istituto scolastico siciliano, deve farci riflettere, colleghi, su quello che può accadere agli inconsapevoli cittadini. Spetta al Ministero valutare se nella conduzione del concorso possano esserci stati errori o disattenzioni. Coloro che sono stati oggetto di questa ingiustizia hanno la necessità di sapere che c'è chi, operando nelle Aule parlamentari, dopo aver preso atto della verità, ridà loro fiducia nelle istituzioni.

Il concorso è stato annullato dalla magistratura amministrativa. Certamente non compete al Governo entrare nel merito della bontà della decisione. La soluzione che abbiamo proposto serve ad assicurare la continuità didattica in una Regione importante come la Sicilia. Come ho già detto in Commissione, posso solo assicurare

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.3, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.5».

GIAMBRONE *(IdV)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervenendo in dichiarazione di voto sull'Atto Senato n. 1929, in materia di concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, annuncio fin da adesso il voto favorevole del mio Gruppo. Vorrei cominciare, signor Presidente, facendo riferimento al commento del ministro Gelmini in occasione di un convegno proprio su questo tema. Il Ministro ha «Abbiamo due doveri: tener conto di un pronunciamento del Consiglio di Stato, che è chiaro, e, allo stesso tempo, accogliere la richiesta del Quirinale, che ha premuto perché si predisponesse un decreto autonomo». È esattamente quello che avevamo chiesto noi, signor Presidente, nella trattazione dello scorso decreto salva-precari. Certamente, le parole del Ministro sembrano molto caute e responsabili e tendono a mettere una toppa ad una situazione partita male finita, a nostro avviso, peggio. Ancora una volta, si è costretti ad operare attraverso una legislazione di copertura per rimediare ad anomalie. Il nostro, così come anticipato, sarà un voto favorevole che scaturisce da alcune considerazioni. Si tratta di un provvedimento che, una volta estrapolato dal decreto salva-precari, consente una disamina approfondita e serena di una questione assai complessa, che non trascuri i principi, per noi irrinunciabili, di rispetto della legalità e l'esigenza di adottare provvedimenti in maniera non frettolosa, né approssimativa. Vorrei ricordare che il concorso dei presidi in Sicilia è stato ritenuto illegittimo dopo un ricorso per procedure scorrette riguardo ad alcune correzioni di elaborati. Successivamente, nel decreto salva-precari (e voglio ricordare, signor Presidente, che proprio questo tiene aperta una ferita profonda sul futuro lavorativo di tantissimi insegnanti), con un colpo di mano, si è cercato di introdurre, attraverso i commi 4-*septies* e 4-*octies*, una minisanatoria, noi ci siamo opposti in Commissione ed in Aula. Non di altro, infatti, si è trattato quando si diceva che «l'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio». Immediatamente, come partito dell'Italia dei Valori denunciammo l'incostituzionalità di questo provvedimento e presentammo un'apposita questione pregiudiziale di costituzionalità, denunciando la nostra non condivisione di emendamenti che, a nostro avviso, apparivano come una scorrettezza da parte dei colleghi proponenti per inserire una norma a tutela di un concorso dichiarato nullo in un decreto che invece, sotto mentite spoglie, si proponeva come nobile scopo quello di salvare i docenti precari dopo la scure Tremonti-Gelmini. A noi questa operazione è sembrata una mancanza di rispetto nei confronti dei professori che legittimamente sono inseriti nelle graduatorie, come si suol dire di questi tempi, senza se e senza ma: la loro posizione è limpida e frutto di regolari abilitazioni ministeriali. Ora i fatti ci hanno dato ragione perché la norma è stata cancellata da un decreto *ad hoc* per evitare conflitti fra poteri e sanare una macroscopica incongruenza normativa. Anche il presidente Napolitano si era espresso in tal senso e aveva sollecitato una revisione del decreto, altrimenti non avrebbe apposto la sua firma. In Sicilia i presidi coinvolti sono circa 420 e certamente un'improvvisa vacanza di posto potrebbe mettere a rischio il normale svolgimento delle attività didattiche, con enormi ricadute sulla qualità scolastica. Noi siamo consapevoli dei gravi disagi che sta attraversando la scuola e la recentissima bocciatura del Consiglio di Stato sul riordino della scuola superiore dovrebbe far riflettere tutti noi su queste riforme calate dall'alto, senza interpellare il termometro della scuola, cioè gli insegnanti, e senza il coinvolgimento delle famiglie. Insomma, non si può continuare con queste operazioni di chirurgia fiscale, anche perché vorrei sottolineare una notizia che probabilmente sta passando inosservata, ma che per il futuro del nostro Paese è molto più importante dei recentissimi fatti di cronaca: il nostro debito pubblico ha toccato, in questo mese, un nuovo record negativo; mai è stato così alto. Ci chiediamo allora come mai, malgrado i risparmi che hanno sacrificato il posto di lavoro di centinaia di persone, il debito dello Stato continui a salire: qualcuno dovrà pure spiegarcelo. In considerazione di tutti questi fatti, siamo favorevoli alla soluzione transitoria adottata dal Governo di concerto con i sindacati, cioè di mantenere in questo momento i presidi nelle loro funzioni e nelle loro sedi fino all'espletamento di una nuova procedura concorsuale che - lo vogliamo dire con grande chiarezza, signor Sottosegretario

addivenire alla interruzione di un servizio pubblico, privando circa un terzo delle scuole siciliane di risorse e competenze maturate grazie ad un lungo e articolato percorso e messe alla prova sul campo senza demerito, spesso proprio nelle sedi più disagiate e a rischio di fenomeni di devianza sociale e deprivazione culturale. di espletare immediatamente un nuovo concorso, che tenga conto di chi è stato anche escluso ingiustamente, al fine di ripristinare la legalità. È questo che le chiediamo, signor Sottosegretario, e mi pare che il suo impegno vada proprio in questa direzione. Ovviamente, fra quei presidi ritenuti idonei non tutti possono essere riconosciuti come falsi vincitori, ma in questa situazione falsata già dall'inizio delle procedure concorsuali è molto difficile scindere il grano dal miglio. che noi vogliamo dire con molta chiarezza che voteremo a favore di questo provvedimento. Mi pare di poter dire che da parte del Governo vi sia la volontà ripetere immediatamente il concorso, per ripristinare le condizioni di legalità che abbiamo chiesto con grande forza durante la trattazione del provvedimento salva-precari, esigenza emersa anche oggi in Commissione, dove c'è stato un dibattito assolutamente importante.

la potremmo configurare come una sorta di caso di scuola, perché è una vicenda stranissima che inizia addirittura nel 2001 e che è connotata da una serie di disparità: disparità di

- stranissima alla luce della vicenda allucinante che stiamo affrontando con questo provvedimento - al minimo a cui il cittadino italiano si può affidare, cioè alla certezza del diritto. Nella realtà, di certezza del diritto in tutta questa vicenda drammatica, in fin dei conti non c'è assolutamente nulla, tant'è vero che nel tempo molti di noi hanno affrontato la situazione con una serie di interrogazioni alle quali pure bisogna

quanto effettivamente di giustizia si possa parlare in questo momento, allorquando, con un intervento del genere, il Consiglio di giustizia amministrativa

Soltanto i dirigenti scolastici siciliani non hanno questo tipo di certezza e vivono ancora in uno stato di precarietà che non dà sicurezza né a loro, né alle loro famiglie, né alle famiglie dei docenti, né alle famiglie degli studenti e, quindi, lascia tutti

di questo provvedimento, ma le assicuro che votiamo con molta amarezza per come sono andate le cose e per una situazione che ci auguriamo non si ripeta mai più in futuro, perché la gente di tutto ha bisogno

sburocratizzare e ad essere chiari e trasparenti; questa vicenda invece ci mostra quanto la burocrazia sia eccessivamente intervenuta e quanto poco trasparente sia stato questo concorso.

il comma 4-*quinquiesdecies* intendeva sanare una serie di anomalie che si riferiscono al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con decreto dirigenziale del 22 Partendo dalle modalità di nomina della commissione esaminatrice, alcuni ricorrenti hanno contestato le modalità con le quali si era proceduto alla correzione degli elaborati scritti, che in alcuni casi avevano prodotto risultati discutibili, attribuendo punteggi elevati a elaborati che contenevano errori ortografici, con correzioni effettuate anche alla velocità di otto facciate in 120 secondi, in pratica 15 secondi a facciata. Dopo i ricorsi presentati dai predetti candidati con i quali si chiedeva «l'annullamento, previa sospensione, della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute al citato corso-concorso selettivo», il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, chiamato a decidere in appello rispetto alla decisione del TAR della Sicilia, che aveva respinto il ricorso principale dichiarandolo inammissibile, ha deciso invece di accogliere il ricorso, emettendo al riguardo ben due sentenze. Nel dispositivo, esaminando i motivi del ricorso in primo grado, si afferma che il collegio ritiene fondato il secondo motivo riproposto, anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. A questo punto si apre uno scenario del tutto nuovo. Non solo, ma si aprono nuovi scenari anche per i partecipanti delle altre Regioni, dove vi sono ancora ricorsi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato per situazioni analoghe a quelle che hanno trovato accoglimento dinanzi all'organo di giustizia amministrativa della Regione Siciliana. Sembra che l'Avvocatura abbia deciso di rinnovare le prove concorsuali. La norma in commento salvaguarderebbe la posizione dei vincitori e degli idonei al predetto concorso, che non dovrebbero sostenere le prove previste dal nuovo regolamento per il reclutamento dei dirigenti, basato sulla selezione per merito (preselezione, concorso basato su due prove scritte e una prova orale, esperienza di almeno 5 anni nel settore e così via). La sentenza 10 novembre 2009, n. 1065 intervenuta mentre era in corso l'*iter* parlamentare del decreto-legge n. 134 del 2009 - ha condotto il Consiglio di giustizia amministrativa a dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine è stato posto un termine di 60 giorni dalla notifica della decisione, con riserva di nomina del commissario *ad acta* ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine. Qualora la suddetta sanatoria legislativa fosse stata approvata, si sarebbe determinato uno scioglimento positivo della riserva operata dalla decisione di merito assunta in sede giurisdizionale così come, nel caso di specie, in ossequio al principio dello *ius superveniens*, in presenza dei predetti contenziosi amministrativi o giurisdizionali si sarebbero fatti cessare i motivi del contendere. Quindi, plaudiamo alla decisione del presidente Napolitano di far espungere questa norma dal decreto-legge n. 134 del 2009, comprendendo tuttavia la necessità di mantenere, in via transitoria, i 378 dirigenti scolastici in parola, onde salvaguardare gli interessi degli istituti scolastici interessati, evitando così di rendere nulli tutti gli atti di gestione posti in essere dai predetti dirigenti. Per questi motivi la Lega Nord esprimerà un voto favorevole.

è doverosa non solo perché rimanga agli atti, ma perché stiamo parlando di un argomento di grandissimo rilievo dal punto di vista istituzionale ed umano.

responsabilità di rilievo nei confronti degli studenti, delle loro famiglie e in genere del futuro di quei ragazzi. Rivolgiamo il nostro grazie ai dirigenti scolastici e agli insegnanti della Sicilia, e agli insegnanti della Sicilia, perché stanno interpretando il loro ruolo a prescindere dalle imprecisioni, addirittura dagli errori di carattere metodologico che hanno inficiato un concorso e lo hanno reso nullo. I miei colleghi sono entrati molto nel merito, anche dal punto di vista giuridico, raccontando fasi che hanno riguardato sia la legislazione sia la giurisprudenza. A me compete solo ricordare perché anche noi voteremo

riguardano gli studenti e i docenti dei singoli istituti e abbiamo bisogno che tutti questi atti vengano considerati assunti

avrebbero potuto essere docenti incaricati di quella funzione. Pertanto, quando si chiede che il 31 agosto cadano dalla funzione, si mette nella condizione di moltissimi altri dirigenti scolastici che non sono vincitori di concorso, non occupano una sede di ruolo, ma hanno soltanto una funzione con un'indennità.

e di regole. Il nostro partito su alcune parole vuole fondare un modo diverso di rapportarsi anche con la maggioranza, affinché si realizzi un linguaggio comune che ci metta nella condizione della mitezza del confronto. Questi dirigenti scolastici sono vittime di un abuso burocratico. Il presidente di una commissione, a suo tempo, aveva deciso lui come interpretare

il dirigente regionale è vivo e vegeto. Si può chiedere al Governo e al Ministero di vigilare, di saper esprimere un giudizio e di prendere le conseguenti iniziative riguardo a dirigenti di così elevato grado che dovrebbero saper interpretare funzioni, ruolo e responsabilità? Sottosegretario, noi ci fidiamo: questa sera il nostro voto su tale decreto‑legge diventa - ahimè - perfino un voto di fiducia al Governo, nel senso che ci fidiamo della tempestività dell'organizzazione di un nuovo concorso.

a un concorso; per dare continuità didattica (tuttavia, i miei colleghi hanno già spiegato - ahimè - quanta continuità didattica abbiamo perso quest'anno e l'anno scorso con i provvedimenti Tremonti-Gelmini); infine, perché credo che il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, anche nel dispositivo della sentenza, abbia chiesto immediata attuazione, espletamento e conclusione entro tempi certi del concorso.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, innanzitutto mi preme chiedere umilmente scusa alla senatrice Adamo per averla interrotta in malo modo; non me ne voglia. So benissimo che la legislazione scolastica non è semplice, ma è molto complicata e non sempre si può essere a conoscenza delle cose.

hanno avuto in prova la loro prima presidenza; hanno superato il periodo di prova e sono diventati a tutti gli effetti presidi, come gli altri. All'improvviso arriva una sentenza

Noi dobbiamo applicare le sentenze. Il Paese segue le regole, giustamente, ma pensate al danno subito da questi presidi che, a loro insaputa, hanno partecipato a un concorso che alla fine è risultato nullo, perché un presidente di commissione contemporaneamente partecipava alla commissione e ad una sottocommissione.

a loro, agli esclusi e a tutti gli altri che vorranno parteciparvi, come a dire che quel concorso è carta straccia. Ebbene, signor Presidente, queste persone, questi cittadini italiani, una volta vinto il concorso e diventati dirigenti, hanno sicuramente pensato ad una prospettiva di vita diversa da prima; hanno preso impegni (è normale), ed oggi si ritrovano

ma non avrebbero ritrovato nemmeno il posto da professori, perché nel frattempo, in questi tre anni, il loro posto è stato occupato da altri. Probabilmente, sarebbero stati messi a disposizione delle scuole o della stessa scuola come supplenti.

presidente di commissione che, tra l'altro, era responsabile della Corte dei conti, era quindi un uomo di legge e non poteva non sapere.

Quella di aver studiato, di aver superato una prova scritta, di aver superato una prova orale e di aver vinto un concorso? È questa una colpa? Ebbene, un Parlamento serio non avrebbe varato questo provvedimento. Un Parlamento serio avrebbe sanato questa situazione. Questa non è una sanatoria, è una burla, perché se io fossi nei panni loro farei un ricorso al direttore generale della Regione Siciliana e al Ministero per danni. Questo farei e probabilmente molti di loro lo faranno, con aggravio di spesa - questo sì notevole - per

DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 Il relatore, senatore Di Girolamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi il provvedimento in titolo concerne l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra Italia e Norvegia. I due Stati si obbligano reciprocamente a fornirsi, su richiesta ovvero spontaneamente, assistenza e cooperazione, mediante le Autorità doganali, per dare completa attuazione alla legislazione doganale e realizzare un'azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni, con l'ulteriore vantaggio della trasparenza dell'interscambio commerciale. Quanto ai contenuti, l'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed un Allegato: l'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 indica il campo di applicazione ed individua le amministrazioni doganali come autorità competenti all'applicazione. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, di informazioni e documenti, elencando casi e finalità. L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali sulla legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. L'articolo 6 prevede lo scambio d'informazioni tra le amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 7 impegna le amministrazioni doganali alla sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che possano essere coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 9 dispone tra le amministrazioni doganali una mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti anche di sequestro, blocco e confisca dei beni e disporre dei beni confiscati in applicazione dell'Accordo. L'articolo 10 individua i casi di assistenza tecnica e l'articolo 11 disciplina il recupero crediti, mentre l'articolo 15 obbliga ciascuna amministrazione doganale, su richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. L'articolo 17 regola lo scambio di dati personali secondo il livello di tutela degli stessi e l'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese e l'articolo 21 detta le procedure di attuazione dell'Accordo, istituendo una commissione mista per l'esame delle questioni connesse alla cooperazione e la mutua assistenza. L'articolo 23 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo, l'articolo 24 ne disciplina l'entrata in vigore, l'articolo 25 la durata e la denuncia e l'articolo 26 il riesame. Quanto al disegno di legge, ricordo che esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in circa 28.000 euro annui. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

sono le ore 19,45 di una seduta al cui ordine del giorno non erano previsti questi tre provvedimenti, per i quali, ricordo, avrei promesso la richiesta di voto elettronico o addirittura - oggi sarebbe particolarmente significativo - la verifica del numero legale, perché si tratta di Accordi internazionali, tra i quali c'è anche un Trattato. Sappiamo che il diritto internazionale ha suprazia

Oggi, forse facendo un rapido giro di Aula, grazie al Gruppo della Lega in modo particolare, si potrebbe arrivare, al limite, ad un risicatissimo numero legale MONTI *(LNP)*. Noi

di iscrizioni a parlare confezionate in cinque minuti. Quando lei, signor Presidente, ha sospeso la seduta per cinque minuti per far distribuire questi documenti - e ringrazio gli Uffici per la solerzia con cui ci sono stati forniti avrebbe anche sperato nell'annuncio della presenza in Aula di un rappresentante del Ministero degli esteri. Certo, il Governo è rappresentato, ma non c'è chi ha seguito in Commissione un *iter* che sicuramente non ha presentato alcun tipo di problema, anche se forse sul Trattato che sarete chiamati a ratificare, in mia assenza, più avanti, riguardo il trasferimento il trasferimento di persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana si potrebbe avere da eccepire circa la qualità delle carceri dell'isola caraibica. carceri dell'isola caraibica. Quindi, auguro al rappresentante del Governo di aver ricevuto, almeno lui, per tempo delle carte e di poter dare un parere articolato relativamente a questi tre provvedimenti. Questo modo di fare - ripeto, io non partecipo al dibattito, ma è l'ultima volta che non chiedo o il numero legale o il voto elettronico - fa sì che il nostro Paese continui a ratificare Trattati internazionali di grande importanza, e me ne vengono in mente almeno due, uno sulla tortura e l'altro sulla creazione della Corte penale internazionale però non è stato ancora ratificato - senza poi prendere alcuna delle misure necessarie per includere le norme del documento in questione all'interno del nostro sistema nazionale. La Corte penale internazionale è un'ottima istituzione, ma non vede l'Italia tra i Paesi che hanno adeguato il proprio ordinamento nazionale in modo da potervi collaborare in maniera efficace. Voglio sapere se un domani diremmo no alla presenza sul suolo patrio di Omar Al-Bashir qualora dovesse essere invitato ad un'altra riunione della FAO o di altre agenzie

malgrado abbiamo presentato più proposte di legge e anche emendamenti all'interno del pacchetto sicurezza, per includere finalmente il reato della tortura, per come è articolato all'interno della Convenzione, nel nostro codice penale, c'è stato prima detto di no

alle ore 19,49, è l'ultima volta che quest'Aula licenzierà un Trattato internazionale senza un voto elettronico.

Signor Presidente, per quanto riguarda le osservazioni circa la rappresentanza del Governo, volevo informare il senatore Perduca che ho avuto l'onore ed il favore di essere parlamentare europeo per nove anni,

l'Accordo è finalizzato ad istituire una migliore collaborazione nel campo giudiziario tra i due Paesi, considerando altresì che nell'ambito degli accordi bilaterali la materia riveste particolare delicatezza, stante la situazione delle carceri domenicane; soprattutto sul trasferimento delle persone condannate risponde quindi ad esigenze umanitarie e favorisce il trascorrere della pena detentiva nel Paese di cittadinanza, favorendone il reinserimento, allo scadere della condanna. Nei contenuti l'Accordo prescrive che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire - conformemente agli accordi internazionali in materia - ad alcune condizioni: che la sentenza di condanna sia passata in giudicato; che la parte della condanna ancora da espiare sia almeno di un anno; che l'infrazione penale sia considerata tale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito; che lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Inoltre, viene stabilito che il condannato, cui può essere applicato il Trattato e che faccia richiesta di trasferimento, deve dare il consenso volontariamente con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti autorità dello Stato di condanna. Per l'adozione della relativa decisione, le autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine. La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi. Le spese derivanti dall'applicazione di questo Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne quelle verificatesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Quanto al disegno di legge, ricordo che si compone delle consueti disposizioni di esecuzione della ratifica,

Signor Presidente, l'Accordo è finalizzato ad istituire una migliore collaborazione nel campo giudiziario tra i due Paesi, considerando altresì che nell'ambito degli accordi bilaterali la materia riveste particolare delicatezza, stante la situazione delle carceri domenicane; soprattutto l'Accordo risponde ad esigenze umanitarie. Pertanto, il Governo auspica la celere ratifica dell'Accordo.

L'Accordo prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, creando il quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Le Le amministrazioni coinvolte sono le amministrazioni nazionali del turismo dei due Paesi. Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo riguardano la collaborazione nelle attività formative settoriali; gli scambi di informazione, di materiale turistico

per segnalare all'Aula la preoccupazione per un clima che si sta effettivamente avvelenando e che sta assumendo toni che rischiano di tornare ad essere quelli sciagurati degli anni Settanta. Nel volantino di rivendicazione di legge testualmente che si tratta di un "attacco ad un avamposto del dominio, dove si formano i nuovi strumenti ed apparati del capitale, dove si affilano le armi che taglieranno la gola agli sfruttati". Al di là del fatto che si tratta fortunatamente di un episodio che non ha prodotto particolari danni, preoccupa questo clima, che ricorda troppo da vicino il clima di scontro

la mano sulla coscienza per riportare il dialogo a termini urbani e contenuti. *(Applausi